verifica del numero legale,

mentre tentano di sfuggire ad una vita di stenti e di miseria ripropongono in tutta la loro dolente drammaticità il tema dell'immigrazione clandestina. Il primo pensiero non può non essere rivolto con forte solidarietà umana alle vittime e ai loro familiari. Ad esso va aggiunto il ringraziamento per tutti coloro - militari, civili ed istituzioni pubbliche - che si prodigano senza sosta nelle operazioni di soccorso. È ormai a tutti evidente che questo problema drammatico va risolto non in maniera isolata, ma con un'azione concertata che veda tutte le Nazioni europee farsi carico di una questione epocale e le Nazioni africane e degli altri Paesi da cui questi infelici provengono coinvolte nell'opera di assistenza e prevenzione. Su questo il nostro Parlamento è chiamato a riflettere, ma ora è il momento della consapevolezza e della solidarietà. Nel ricordo di queste vittime, ma anche - con drammatica coincidenza - nel ricordo delle sei vittime anch'esse morte in Sicilia per un infortunio sul lavoro, delle quali proprio oggi si svolgono i funerali, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

espressioni di cordoglio e di lutto per la serie, ormai interminabile, di tragedie legate al grande fenomeno delle immigrazioni. Ritengo

il Partito Democratico non condivide. Ma il tema della sicurezza è di grandissima importanza per il nostro Paese, per l'Europa e per tutto il mondo.

a venire in Parlamento ad esporre una strategia di prevenzione, rispetto alla necessità di contenere questa immane tragedia legata alle immigrazioni. *(Applausi finestra"). La Presidenza si farà carico della sua richiesta, invitando il Governo a riferire al più presto in quest'Aula sulle linee guida della sua politica di prevenzione sul tema, a noi tanto caro, degli infortuni sul lavoro.

Si tratta di questioni che attengono ai rapporti tra i diversi poteri dello Stato, ad un assetto, ad un equilibrio o ad un riequilibrio tra i poteri dello Stato. Si parla di norme che tenderebbero a bloccare i processi e a garantire l'immunità per le alte cariche dello Stato.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che l'epistolario intercorso tra il presidente del Consiglio Berlusconi e lei, che ricopre la carica di Presidente di questa Assemblea e che è la seconda autorità dello Stato, non possa essere considerato un epistolario privato,

Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento del Senato, vorrei pregarla di valutare quanto prima la possibilità di calendarizzare la mozione n. 1, quella, cioè, relativa alla problematica dello scioglimento del Consiglio regionale della Campania. La situazione da noi è tragica. Continua la farsa di un'amministrazione regionale incapace di governare. È di ieri un'intervista rilasciata a «Il Mattino»

dichiarando che si sta preparando un'altra tornata di contributi a pioggia, quindi di sperpero dei fondi europei. Pertanto, signor Presidente, visto che i termini sono già scaduti da qualche settimana, la pregherei

di dare lettura di questa lettera nel momento proceduralmente corretto, una volta incardinato l'argomento che stiamo per discutere. Quindi, immediatamente dopo la replica

dal momento che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento ammette la possibilità di presentare questioni pregiudiziali anche successivamente all'avvio della discussione e che tale discussione non può certo considerarsi conclusa perché i relatori non hanno replicato, ci appare necessario presentare una questione pregiudiziale in relazione all'emergere di nuovi elementi che modificano radicalmente il senso complessivo del disegno di legge di conversione. La lettera inviata dal presidente Berlusconi al presidente Schifani indica con chiarezza che gli emendamenti presentati in Assemblea dai relatori, senza alcun preventivo vaglio delle Commissioni referenti di cui i relatori sono altresì Presidenti, devono ritenersi direttamente riconducibili al Governo e, più specificamente, al Presidente del Consiglio scrivente. Essi dovrebbero essere dichiarati inammissibili ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento, secondo gli stretti canoni interpretativi contenuti nel parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984. Infatti, è lo stesso Presidente del Consiglio che, nella medesima lettera, rivela come la norma introdotta per via emendativa sia applicabile ad un processo in corso nei suoi confronti, con ciò rendendo evidente che la data del 30 giugno 2002 non sia legata a novità normative oggettive ma che fotografi un caso particolare. Per di più, la medesima missiva spiega che la sospensione dei processi costituisce l'anticipazione di una successiva riforma costituzionale per tutelare le più alte cariche dello Stato. Per dì più ancora, motivando congiuntamente l'emendamento e la ricusazione di un giudice in un determinato processo, l'eventuale voto favorevole a tale emendamento si trasformerebbe anche in una espressione di consenso a questa ricusazione. In tal senso, la lettera andrebbe considerata irricevibile almeno in tale parte affinché l'istituzione del Senato non sia accusata di interferire nell'ordine giudiziario. Nel merito dell'emendamento proposto, non può che rilevarsi come non si tratti di norme urgenti in materia di sicurezza pubblica ma di norme relative alla protezione dei titolari *pro tempore* delle più alte cariche istituzionali, pur apparentemente mascherate da norme generali ed astratte, in vista della tutela definitiva offerta dalla annunciata riforma costituzionale che dovrebbe entrare in vigore prima della scadenza dell'anno di sospensione. In secondo luogo, anche ammesso e non concesso che si tratti di emendamenti ammissibili relativamente alla pertinenza, in modo del tutto illegittimo essi inseriscono nuove disposizioni incostituzionali in relazione al principio di uguaglianza, sia per gli imputati sia per coloro che richiedono giustizia, discriminati sulla base di un limite temporale del tutto arbitrario, non giustificato da circostanze oggettive; incostituzionalità che sarebbe superata solo sulla base della forza dei numeri della maggioranza, non disponendo i parlamentari nel nostro Paese di strumenti quali il ricorso preventivo sulla costituzionalità delle leggi di fronte all'organo di giustizia costituzionale. In terzo luogo, gli emendamenti, modificando comunque in modo qualitativo la legge di conversione, al di là degli stessi profili di mancata pertinenza e di incostituzionalità, pongono delicatissimi problemi di rapporto col potere presidenziale di rinvio delle leggi sulla base del vigente articolo 74, il quale prevede esclusivamente il rinvio di un'intera legge e non anche di parti di essa, che invece, ad esempio, l'istituto del *referendum* abrogativo, di cui all'articolo successivo, ammette. La Presidenza della Repubblica, come da anni sottolinea con preoccupazione la dottrina, si trova pertanto di fronte a due alternative, entrambe rigide: rinviare tutta la legge di conversione, dopo aver avallato in origine l'esistenza dei requisiti di necessità e urgenza, o soprassedere del tutto di fronte a dubbi di pertinenza e di costituzionalità. Dal momento che la lettera del presidente Berlusconi assume di fatto la paternità degli emendamenti, è peraltro evidente che l'inserimento a questo punto dell'*iter* è dovuto all'intento di sfuggire al sindacato di costituzionalità sotto i profili, sia del merito sia dei requisiti di necessità e urgenza, tanto da parte della Presidenza della Repubblica, quanto delle Commissioni parlamentari competenti. Per queste ragioni riteniamo necessaria la sospensione dell'esame in Aula di una legge di conversione che ha mutato profondamente natura, da misure per la sicurezza dei cittadini a misure per la messa in sicurezza del Presidente del Consiglio dai giudici, e richiediamo il suo rinvio alle Commissioni referenti a cui è stato arbitrariamente sottratto l'esame di disposizioni così importanti e decisive per la natura del provvedimento.

discussi ed eventualmente posti in votazione. Per quanto attiene alla sua richiesta di pregiudiziale, le significo che la discussione generale è stata dichiarata chiusa, con

È vero che la questione pregiudiziale può essere proposta nei termini e con la scansione temporale prevista dal primo capoverso dell'articolo 93, ma è altrettanto vero, come è stato detto dal collega Ceccanti, che «nel corso della discussione» - così testualmente recita il Regolamento - ed in presenza di nuovi elementi, si può nuovamente proporre una questione pregiudiziale, ovviamente in rapporto a tali nuovi elementi. Lei ha dichiarato, seppur non formalmente, di non ritenere ammissibile, benché il Regolamento l'autorizzi a farla discutere e votare, la questione pregiudiziale proposta in questa fase temporale del procedimento.

ove il Governo o il relatore intendessero presentare una proposta nuova nell'arco di svolgimento dell'*iter* legislativo,

collocare tale proposta esattamente in questa fase, sfuggendo in questo modo a qualunque possibilità, per l'Aula del Senato, di sindacarne la costituzionalità.

La prima richiesta è che questo punto specifico - non so se vi siano precedenti in questo senso - sia sottoposto alla Giunta per il Regolamento perché decida sulla questione

secondo la quale le questioni pregiudiziali non possono essere materia di discussione in ordine agli emendamenti proposti. Io ritengo che il comma 1 dell'articolo 93 del Regolamento assegna a lei, signor Presidente, ampi poteri, qualora fatti nuovi sopravvenuti rendano evidente la necessità di affrontare temi afferenti le pregiudiziali. È un potere affidato alla sua sensibilità e ad una interpretazione dinamica del Regolamento. Abbiamo esaminato le questioni pregiudiziali all'inizio della discussione con un corpo di norme che aveva uno specifico contenuto. Oggi quel corpo di norme è raddoppiato rispetto al contenuto originario.

Si interviene ora in materia di modifica dei compiti del Consiglio superiore della magistratura, di trasferimento di magistrati, di sedi disagiate, di aumento delle piante organiche della magistratura, di norme di attuazione di norme di attuazione del codice di procedura penale e di individuazione di priorità dei processi da celebrare. Si tratta dunque di un complesso di norme che non era stato neanche sfiorato nel corso dell'esame in Commissione. Non è pensabile un'interpretazione restrittiva del Regolamento, che sarebbe preclusiva di tutta la materia - che indubbiamente esiste - di natura costituzionale, cui afferisce questa nuova parte che si intende introdurre con gli emendamenti presentati al decreto-legge in conversione. Quindi, signor la sollecito, facendo appello alla sua sensibilità di giurista, ad interpretare l'articolo 93 nel modo più saggio, cioè nel senso di dare la possibilità alle Commissioni o ai singoli senatori di intervenire sul nuovo corpo proposto, totalmente diverso da quello sinora esaminato. Se quel nuovo corpo proposto offre materia di discussione, per la serietà del nostro ruolo, io ritengo che la sua imparzialità e il suo ruolo *super* *partes* debbano consentirle di appropriarsi sino in fondo del comma 1 dell'articolo 93, che è norma generale, con l'assegnazione dei poteri che riguardano proprio lei e soltanto lei, signor Presidente. Indubbiamente le questioni proposte sono talmente serie

fatto e proposto degli emendamenti che stravolgono il contenuto originario del decreto. Esistono norme di prassi e di correttezza istituzionale che bisogna sempre rispettare: in Commissione

un discorso di correttezza istituzionale, perché non si possono prendere in giro i rappresentanti del popolo invitandoli a non insistere su emendamenti che avrebbero stravolto

la sollecito a ridare al Senato la dignità di esaminare i disegni di legge con la profondità che i contenuti proposti richiedono.

Ci sono questioni, come quella che riguarda il pronunciamento della Commissione affari costituzionali sui requisiti di necessità ed urgenza, quindi sulla costituzionalità

con una certa formulazione, ottiene addirittura l'autorizzazione e la firma del Presidente della Repubblica; per poter subire degli emendamenti

me lo permette, un'altra annotazione velocissima, perché non voglio abusare della sua cortesia, richiamando le parole con cui il nostro Presidente, ancorché relatore del provvedimento, ha presentato il lavoro fatto dalla Commissione, significandone, al di là della divergenza di opinioni, l'impegno e la voglia di trovare, pur nelle differenze che ancora c'erano, dei punti comuni. Com'è possibile che oggi tutto quel lavoro venga vanificato da una procedura che, a mio parere, non solo ai sensi stretti del Regolamento ma a quelli molto più ampi

nella nostra Carta costituzionale. Quando sono stati presentati questi emendamenti, in particolare l'emendamento 2.0.800 ed i successivi, io sono letteralmente saltato sulla sedia, perché c'è stato uno stravolgimento sia dei Regolamenti parlamentari sia della nostra Carta costituzionale. Siamo in fortissimo contrasto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento, con particolare riferimento al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e della separazione e dell'autonomia della magistratura rispetto al potere politico in senso lato, in particolare al Governo ed al Parlamento. Di fronte ad una proposizione in questi termini e in questi modi, aggirando il potere e il dovere di controllo del Presidente della Repubblica, credo che dobbiamo sottoporre in prima battuta a questa Assemblea la questione pregiudiziale relativa all'urgenza e alla necessità e la questione della costituzionalità così come emerge da questa impostazione. Sono troppe e troppo grandi le rotture rispetto all'ordinamento costituzionale per non dover essere segnalate e, di fronte ad una rottura della legalità costituzionale, non possiamo rimanere inerti. È nostro compito e dovere intervenire e chiedere un voto, innanzitutto - come ha chiesto il collega Legnini in prima battuta - sulla ammissibilità

attenzione gli interventi dei senatori dell'opposizione che hanno affrontato alcune tematiche. Vorrei ricordare ai colleghi che è prassi consolidata, senza eccezione alcuna, cioè, nella storia del Senato e di quest'Aula

esaurita la discussione generale. Quindi, la prassi consolidata, ribadisco senza eccezione alcuna, è questa, anche perché confermata dal comma dal comma 7 dell'articolo 93 del Regolamento, che, proprio a conferma dei precedenti, sostiene che «La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti», a proposito di emendamenti citati dall'opposizione. Detto questo, vi sono osservazioni che possono essere meglio sviluppate in Aula nel merito, come quella del collega Casson sugli emendamenti, e vorrei ricordare come la Commissione affari costituzionali è presente attraverso i suoi componenti in quest'Aula e può, in sede di discussione di merito, intervenire e disquisire in fase di esame degli emendamenti sull'eventuale esistenza o meno dei presupposti

in contrasto almeno con le altre che sono state qui riferite dal senatore Legnini rispetto alla proposizione di nuovi argomenti ed elementi.

Incostante, la Presidenza si riserva di sottoporre alla Giunta per il Regolamento le riflessioni introdotte in questo dibattito dal collega Legnini nel momento in cui ve ne saranno i presupposti e le opportunità. Sicuramente sarà fatto. INCOSTANTE *(PD)*.

Ora, io insisto, Presidente, perché al di là del merito, che pure non è di poco conto, noi dovremmo decidere, con il suo aiuto mi auguro, se in della proposta in discussione. E non mi si dica che non è un elemento nuovo la proposizione di una norma che prevede la sospensione dei processi per il Presidente del Consiglio: che cos'altro deve succedere, signor Presidente? Che cosa deve succedere, quali altri elementi nuovi si devono verificare per poter vagliare la costituzionalità di un provvedimento? Si può votare o non si può votare? Noi non le stiamo chiedendo nulla di più. Le stiamo chiedendo di far esprimere i colleghi, con un voto, sulla questione

sapere se in presenza di un fatto nuovo di grande rilevanza, l'Aula del Senato può esprimersi sulla costituzionalità di una proposta che stravolge il provvedimento, come è stato sottolineato dai colleghi. Quindi, io le chiedo di dirci se vuole farci votare o meno. *(Applausi Collega Legnini, per la Presidenza gli emendamenti sono tutti da trattare alla pari, al di là del loro contenuto, perché tendono a modificare i provvedimenti. Ricordo al collega Legnini e all'Aula che non esiste precedente alcuno in relazione all'accettazione di pregiudiziali a discussione generale conclusa.

la Presidenza sta ascoltando con la doverosa attenzione gli interventi di tutti i senatori dell'opposizione, consentendo loro di esprimere tutte le loro argomentatissime motivazioni. Pregherei, però, i colleghi dell'opposizione, di consentire all'Aula,

io appartengo ad una tradizione politica che degli aspetti formali fa anche una questione di sostanza - e nello stesso momento anche con rispetto personale nei suoi confronti.

Da una parte, Presidente, vi è una questione che riguarda la valutazione della ammissibilità di un emendamento in sede di decreto‑legge, e sappiamo perfettamente che si tratta di una questione più volte esaminata con attenzione anche dalla Corte costituzionale; vi è la questione relativa all'attinenza dell'emendamento rispetto alla materia trattata dal decreto-legge. Se si decide di avere un criterio largo sull'ammissibilità di questioni che non sono esattamente e direttamente oggetto dell'esame del decreto-legge, lei capisce perfettamente che si apre un *vulnus* molto delicato anche perché, Presidente, il Regolamento del Senato è particolarmente severo, anche rispetto a quello della Camera, circa la prudenza con cui va trattata tutta la questione relativa ai decreti‑legge. Ad esempio, al Senato, in Commissione affari costituzionali ed eventualmente in Aula, c'è una valutazione molto severa sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. Allora, se da un lato noi consentiamo l'ammissibilità di emendamenti non attinenti e dall'altro, nello stesso identico momento, in Aula piombano emendamenti di questo tipo, senza che la Commissione competente possa esprimersi, lei capisce perfettamente che si apre una questione per la quale alcune iniziative possono in ogni caso venire a modificare rigidamente il percorso preferenziale che viene assegnato ai decreti-legge. Per questa ragione, Presidente, la prego di considerare nella sua complessità la questione, che è troppo delicata per essere guardata con un atteggiamento esclusivamente di riferimento alla prassi in ordine a qual è il momento in cui può essere presentata una questione di legittimità. Il complesso delle questioni va rimesso alla sua personale valutazione e a quella della Giunta per il Regolamento, per cui noi ci permettiamo di insistere che vada considerato anche questo aspetto, che è delicato e centrale per il funzionamento delle nostre Istituzioni. *(Applausi

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito svoltosi la scorsa settimana ha sostanzialmente confermato l'opportunità, oltre che la necessità e l'urgenza, del decreto-legge in conversione. Da tutti gli interventi dei colleghi di maggioranza e, in maniera più articolata e in qualche caso reticente, anche da quelli dell'opposizione, sono emersi con chiarezza due elementi: l'esistenza di un grave disagio ed allarme sociale derivante dalla criminalità diffusa, e il fatto che, specialmente nell'Italia settentrionale, il tipo di reati che contribuisce soprattutto a determinare questa situazione di allarme e di incertezza è commesso prevalentemente da immigrati clandestini e da persone di cittadinanza rumena. Ciò posto, è evidente che le disposizioni dirette da un lato a favorire l'espulsione e l'allontanamento dei soggetti socialmente pericolosi appartenenti a queste categorie, e dall'altro a sottolineare il disvalore della clandestinità come *status* che oggettivamente integra un atteggiamento di ribellione nei confronti del potere sovrano dello Stato - come è stata definita dal senatore Mazzatorta rivestono la caratteristica di provvedimenti diretti a favorire un'immediata riduzione della tensione sociale legata a queste forme di criminalità, che costituisce la *ratio* del provvedimento d'urgenza; si tratta in sostanza di disposizioni - rese, lo voglio ricordare, ancora più efficaci proprio grazie all'accoglimento di emendamenti proposti dall'opposizione che hanno lo scopo di consentire allo Stato di ripristinare la sua capacità di controllo e di contenimento di fenomeni oggettivamente devianti. Alla stessa logica di urgenza, del resto, si ispirano le disposizioni in materia di circolazione stradale, che pure tutti hanno condiviso. Le principali critiche avanzate dall'opposizione nel corso del dibattito in realtà, oltre che vertere sulla questione della legittimità costituzionale dell'aggravante generale introdotta dall'articolo 1, hanno avuto ad oggetto questioni che esulano dal contenuto di un provvedimento di urgenza. Da un lato, infatti, l'opposizione ha rimproverato al Governo di non avere introdotto disposizioni dirette alla repressione di specifiche fattispecie di reato o in qualche caso alla loro creazione *ex novo*, sulle quali evidentemente deve invece svolgersi un confronto approfondito e non dettato da motivazioni di urgenza, dall'altro hanno accusato il Governo di non intervenire sulle cause che determinano la clandestinità e che vengono individuate specialmente in limiti eccessivi all'accesso di lavoratori regolari o alla loro permanenza. Sotto quest'ultimo profilo, se da un lato non c'è dubbio che bisogna ad esempio studiare nuove procedure per rendere meno disagevole il rinnovo del permesso di soggiorno ma evidentemente si tratta di questione che esula totalmente dall'ambito di questo decreto-legge - va peraltro ribadito che questa maggioranza non solo non può convenire sull'idea che il rimedio alla clandestinità possa essere trovato nella eliminazione di quelle regole di accesso la cui violazione determina la clandestinità stessa, ma non può che ribadire il principio che il fenomeno della immigrazione deve essere regolato dallo Stato alla luce delle effettive possibilità di assorbimento degli stranieri da parte della società italiana non solo sotto il profilo economico, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ma anche sotto quello culturale.

prendere atto che esaminiamo un provvedimento sul quale ci siamo ampiamente confrontati in Commissione e in Aula e su cui sono emerse significative convergenze ed anche alcuni temi temi sui quali non siamo riusciti a trovare un accordo che vada al di là di quello della maggioranza parlamentare. Debbo sottolineare, però, che è venuto dall'opposizione sin qui un contributo positivo allo svolgimento del dibattito e che il provvedimento che ci troviamo ad esaminare contiene anche emendamenti (almeno sedici) che sono stati approvati in Commissione con il concorso dell'opposizione ed essendo stati presentati dalla stessa opposizione. opposizione. Nel ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alla discussione generale per il contributo ulteriore che hanno apportato e valutata la fase iniziale del dibattito di questa mattina, che anche gli emendamenti che dovremo esaminare nel corso di questo dibattito, nei modi e nelle forme che il Regolamento prevede e che il Presidente saprà abilmente guidare, possano vertere il merito delle materie che stiamo discutendo stiamo discutendo senza atteggiamenti pregiudiziali e senza investire questioni personali, ma soltanto per valutare quello che si è scritto, quello che si deve approvare, quella che è la via migliore per dare risposta a problemi urgenti nella coscienza e nella vita della nostra società.

necessità e della urgenza, ma ha anche registrato una serie di votazioni unanimi su diversi articoli del decreto-legge. Vi è infatti una percezione, da parte dell'intero Parlamento, del senso di insicurezza che i cittadini avvertono rispetto a quei fenomeni che vengono descritti nella relazione al disegno di legge e che hanno trovato puntuale espressione nelle norme che sono state introdotte all'articolo 1, su suggerimento dell'opposizione. Mi riferisco, in particolare, alle norme che riguardano la falsa attestazione o dichiarazione di un pubblico ufficiale sull'identità e qualità personale proprie e di altri, alle norme sulle fraudolenti alterazioni per impedire l'identificazione o gli accertamenti di qualità personali, alle false dichiarazioni sull'identità personale. Vi è poi una serie di modifiche al testo del decreto-legge, in particolare agli articoli 10, 11 e 12 che sono stati emendati dal Governo con un

vostra attenzione - sul versante della lotta alla mafia, delle misure di prevenzione e dei poteri che vengono attribuiti oltre che ai procuratori distrettuali e al procuratore ordinario, al direttore della Direzione investigativa antimafia.

in una complessiva valutazione dell'intero decreto-legge, per quanto riguarda una calibratura delle sanzioni che sono state corrette in più passaggi del decreto-legge con un contributo determinante dell'opposizione.

da pervenire ad un testo che viene presentato in Aula con il massimo dell'approfondimento e del consenso da parte di tutti. Credo che

che richiamano ulteriori reati di violenza contro le donne e i minori: il Governo condivide pienamente che quei problemi hanno necessità di un intervento legislativo e denunciano una situazione di sofferenza, ma ha

Grazie, in appendice alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritengo sia questo il momento perché la Presidenza dia lettura della lettera ricevuta ieri dal Presidente del Consiglio dei ministri. «Caro Presidente, come Le è noto stamane i relatori Senatori Berselli e Vizzini, hanno presentato al cosiddetto "decreto sicurezza" un emendamento volto a stabilire criteri di priorità per la trattazione dei processi più urgenti e che destano particolare allarme sociale. In tale emendamento si statuisce la assoluta necessità di offrire priorità di trattazione da parte dell'Autorità Giudiziaria ai reati più recenti, anche in relazione alle modifiche operate in tema di giudizio direttissimo e di giudizio immediato. Questa sospensione di un anno consentirà alla magistratura di occuparsi dei reati più urgenti e nel frattempo al Governo e al Parlamento di porre in essere le riforme strutturali necessarie per imprimere una effettiva accelerazione dei processi penali, pur nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali. I miei legali mi hanno informato che tale previsione normativa sarebbe applicabile ad uno fra i molti fantasiosi processi che magistrati di estrema sinistra hanno intentato contro di me per fini di lotta politica. Ho quindi preso visione della situazione processuale ed ho potuto constatare che si tratta dell'ennesimo stupefacente tentativo di un sostituto procuratore milanese di utilizzare la giustizia a fini mediatici e politici, in ciò supportato da un Tribunale anch'esso politicizzato e supinamente adagiato sulla tesi accusatoria. Proprio oggi, infatti, mi è stato reso noto, e ciò sarà oggetto di una mia immediata dichiarazione di ricusazione, che la presidente di tale collegio ha ripetutamente e pubblicamente assunto posizioni di netto e violento contrasto con il Governo che ho avuto l'onore di guidare dal 2001 al 2006, accusandomi espressamente e per iscritto di aver determinato atti legislativi a me favorevoli, che fra l'altro oggi si troverebbe a poter disapplicare. Quindi, ancora una volta, secondo l'opposizione l'emendamento presentato dai due relatori, che è un provvedimento di legge a favore di tutta la collettività e che consentirà di offrire ai cittadini una risposta forte per i reati più gravi e più recenti, non dovrebbe essere approvato solo perché si applicherebbe anche ad un processo nel quale sono ingiustamente e incredibilmente coinvolto.

e migliaia di udienze che mi hanno gravato di enormi costi umani ed economici, che sia indispensabile introdurre anche nel nostro Paese quella norma di civiltà giuridica e di equilibrato assetto dei poteri che tutela le alte cariche dello Stato e degli organi costituzionali,

La informo quindi che proporrò al Consiglio dei Ministri di esprimere parere favorevole sull'emendamento in oggetto e di presentare un disegno di legge per evitare che si possa continuare ad utilizzare la giustizia contro chi è impegnato ai più alti livelli istituzionali nel servizio dello Stato. *F.to.* Silvio Berlusconi».

conoscendola, credo che lei abbia colto la gravità del contenuto della lettera che ci ha testé letto. con la lettura di questa lettera purtroppo la legislatura sta assumendo un profilo molto diverso da quello che aveva all'inizio. Immagino che anche lei avrà colto lo stridente contrasto del contenuto di questa missiva rispetto alle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio,

dialogo e della ricerca di larghe maggioranze sui temi di maggiore delicatezza per il Paese. Questa lettera, viceversa, ci spiega in un modo che definirei sfacciato e spudorato che il Senato della Repubblica è chiamato ad esaminare un emendamento che ha l'obiettivo specifico, denunciato anche dalla data

era forte, che andava a toccare un nervo scoperto ed indicava un'affermazione grave del Presidente del Consiglio; nessuno di noi lo ha sollevato per rispetto istituzionale.

Senatore Zanda, la Presidenza prende atto della sua richiesta di un'ulteriore attribuzione dei tempi prende atto della sua richiesta di un'ulteriore attribuzione dei tempi e si riserva, in relazione all'andamento dei lavori, di prenderla in esame nelle sedi e nelle forme più opportune. Sarà fatto senz'altro. GARRAFFA

Paese si renda conto della gravità e della delicatezza del momento. della obbligatorietà dell'azione penale, che si è tradotta nel nostro Paese in arbitrarietà dell'azione penale. Ma non è così che ci si arriva, cari colleghi. Una cosa l'ha detta, il Presidente del Consiglio,

Presidente, la lettera che lei ha letto pone una pietra tombale sull'esito di questa legislatura

Potete anche governare o "sgovernare" per cinque anni, ma è il Paese che entra ormai in sofferenza democratica. *(Applausi Mi rendo conto che la *claque* deve applaudire, ma vorrei finire il mio ragionamento. *(Commenti)*.

ma quanto dolce lo verifichiamo, perché sono le garanzie che vengono meno. È evidente che stiamo parlando di un altro provvedimento e se è un altro provvedimento la tempistica con cui deve essere esaminato deve essere la più congrua possibile, signor Presidente. Lei non può dirci sempre «no, no, no», «vedremo», «sapremo». È stato chiesto

i colleghi Zanda e Belisario. Al collega Belisario rispondo garbatamente e con serenità dicendo che la richiesta di un'ulteriore attribuzione di tempi verrà esaminata dalla Presidenza

a tanti autorevoli colleghi della maggioranza i quali sanno benissimo che, al di là del dialogo istituzionale, del *fair play* istituzionale e anche della possibilità di confrontarsi seriamente - così come è stato detto sui problemi urgenti ed immediati rispetto all'agenda del Paese, esiste anche una questione di fondo: il rispetto di alcune regole che ci tengono insieme, le regole democratiche e costituzionali. Tanti autorevoli colleghi del centrodestra sanno che con la presentazione di questo emendamento annunciato

altrettanti comportamenti del tutto fuori dalle regole prefissate. Noi un giorno potremmo infatti avere un altro emendamento che decide di sospendere i processi, per altre questioni, su altre materie. Stiamo stravolgendo alcune regole degli equilibri istituzionali della separazione dei poteri. Come ha detto la senatrice Bonino, si può discutere su tutto e la maggioranza ha l'onere - direi, - di impostare una discussione, di avanzare una proposta su riforme dell'ordinamento giudiziario, su riforme costituzionali, ma tutto questo non si può fare con emendamenti che arrivano alla chetichella, all'ultimo momento, dopo che

facendo di questo provvedimento, attraverso questi articoli, qualcosa di ben diverso e che incide su altre materie. Signor Presidente, siamo molto preoccupati. Avevamo apprezzato il tono del Presidente del Consiglio, pur consapevoli che ci saremmo divisi su tante e tante questioni; avevamo apprezzato anche lo stile di inizio di questa legislatura, peraltro da noi sollecitato anche in campagna elettorale. Con questa lettera, signor Presidente, davvero...

parli dei suoi legali e dei suoi processi, facendo riferimento all'Aula del Senato, al Parlamento italiano, ai problemi del Paese. Prego davvero di riflettere e suggerisco di ascoltare le proposte prudenti, che tanti hanno avanzato, di convocare la Conferenza dei Capigruppo.

Signor Presidente, i colleghi Zanda, Belisario e Bonino hanno già detto molto bene del carattere inaudito dell'emendamento di fronte al quale ci troviamo. E la prima volta che in questo Parlamento il Presidente del Consiglio ha l'impudenza

«ai fini della necessaria armonizzazione e messa a punto delle prassi seguite nei due rami del Parlamento per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti in sede di conversione in legge dei decreti-legge». Siamo esattamente in questo caso. «L'adozione di criteri rigorosi, diretti ad evitare sostanziali modificazioni del contenuto dei decreti-legge, è infatti indispensabile» - diceva il Quirinale quel giorno - «perché sia garantito in tutte le fasi del procedimento Signor Presidente, siamo di fronte ad una violazione palese di questo di questo precetto, di questa indicazione del Presidente della Repubblica. Come è stato detto nel corso degli altri interventi che si sono succeduti, lei come Presidente di questo Senato, seconda carica della Repubblica, ha il dovere di prendere in considerazione queste preoccupazioni e indicazioni. Se non lo vuole fare per quanto le stiamo dicendo in questa sede, lo faccia per il rispetto dovuto da quest'Aula parlamentare alla Presidenza della Repubblica.

presentazione di un emendamento che riguarda tutti i processi. Qui si propone addirittura di sospendere tutti i processi, di negare quindi giustizia a tutti coloro che l'aspettano. Considerato che è noto che i nostri processi penali già durano all'infinito, mi sono meravigliato, quando si è fatto

un provvedimento che tende a negare giustizia a tutti per agevolare il Presidente del Consiglio.

che prima siano passati al vaglio né del Presidente della Repubblica, né delle Commissioni di merito competenti. Ora si aggiunge anche questo emendamento sul concorso delle Forze armate nel controllo del territorio.

riscontri i suddetti requisiti di necessità e urgenza; in sede di conversione del decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 77 deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso,

che le nostre proposte di prevedere delle fattispecie di reato contro la grande criminalità organizzata non sono urgenti, mentre lo sono soltanto

*(PD)*. Signor Presidente, stiamo assistendo ad un cambiamento anche semantico: necessità ed urgenza si sono ormai sistematicamente tradotti in emergenza. Questo è un Governo che vuole andare avanti per i prossimi cinque anni ponendo una serie di emergenze: rifiuti, intercettazioni, *caveat*, infrastrutture, energia e sicurezza. Siamo stati bombardati dal primo giorno con una serie di emergenze fino ad aver scoperto oggi - e mi pare che la lettera del presidente del Consiglio Berlusconi in qualche modo lo certifichi - la vera emergenza, che è stata inclusa nel quadro di un problema che affronta tutta la società, quello dell'amministrazione della giustizia, che viene chiamata vera e propria emergenza sociale. Ebbene, la senatrice Bonino ha chiaramente esplicitato che in questo Paese, in effetti, un'emergenza sociale relativamente all'amministrazione della giustizia esiste, di sistematica e quotidiana violazione dei diritti umani dei cittadini italiani. Non è possibile che in un Paese esistano dieci milioni di processi sospesi, divisi tra civili e penali, che si protraggono per dieci anni. Quindi, chiunque qui dentro ha sicuramente un problema con la giustizia. Riteniamo che si debba non passare all'esame di questo tipo di misure, proprio perché se c'è un'emergenza - e questa c'è - essa va affrontata in altro modo. Mi unisco quindi alla richiesta dei colleghi senatori del Gruppo del PD,

noi radicali siamo da sempre stati attenti ed abbiamo più volte sollecitato, anche con *referendum* e proposte di legge di iniziativa popolare, la riforma della giustizia e anche la non obbligatorietà

facendo decreti che parlano di altro e poi intervengono su altre materie? I decreti devono avere presupposti di necessità ed urgenza; ma di quale necessità ed urgenza stiamo parlando,

nuova finestra"). In relazione alle numerose richieste di intervento, anticipo all'Aula, anche per meglio e correttamente disciplinare l'andamento dei lavori, che è intenzione della Presidenza consentire a chiunque ne faccia richiesta di intervenire,

ritenesse che un'iniziativa di questo genere non avrebbe determinato un grave strappo a tale clima? Questa è la domanda.

Ad un certo punto diventa più importante la vicenda personale dei destini di una Nazione, perché lei sa quanto questo Paese abbia bisogno di dialogo, di volontà di convergere sui grandi temi di interesse comune. Davanti a questa esigenza - invocata anche da grandi agenzie di formazione e da grandi istituzioni morali di questo Paese - la risposta qual è? Mettere al primo posto i destini personali e posporre quelli della Nazione; tutto questo in un'Aula nella quale ci sono esponenti storici di questo Paese che hanno dimostrato personalmente di avere fiducia nella giustizia, nella magistratura e nelle istituzioni:

questo è un motivo in più per chiederle di riunire la Conferenza dei Capigruppo; non c'è niente di male nel cercare di riorganizzare i lavori insieme, perché dobbiamo comunque lavorare assieme e certamente a me dispiace poter parlare più di altri che magari hanno ragioni migliori.

sera e, in particolare, alla senatrice Poli Bortone, al senatore Benedetti Valentini e non vorrei dimenticarne altri, che, in un'Aula piena solamente di esponenti

Inoltre, le dico che questa lettera, a mio avviso, lede prima di tutto l'immagine e il ruolo della Presidenza del Senato e anche dei relatori Vizzini e Berselli, i quali hanno svolto un lavoro che possiamo anche non apprezzare politicamente, ma che comunque è stato portato in quest'Aula che viene completamente asfaltato da questa lettera inviata dal Presidente del Consiglio. Vi invito, cari amici della maggioranza, a tener conto del fatto che alcune scelte

con il suo atteggiamento sta assumendosi una responsabilità grave di non sospendere i lavori per riunire i Capigruppo o, come ha detto il collega Casson, per riunire la la Giunta per il Regolamento. Abbiamo a che fare con una lettera che ha totalmente stravolto il senso di democrazia. Sappiamo che il Presidente del Consiglio è allergico, come dice il nostro presidente Di Pietro e come diciamo noi, allo Stato di diritto. Dunque non ci siamo, signor Presidente, se continuiamo così. Non siamo nello Stato di diritto ma in un'altra situazione: siamo ancora una volta di fronte al tentativo del principe, questa volta collegiale,

Presidente, lei ci letto una lettera delicatissima e ne è cosciente. Lei è il Presidente del Senato e deve ristabilirne la dignità. I primi passi della lettera che ci ha letto parlano di un cittadino che si rivolge ai propri avvocati per chiedere se gli emendamenti depositati dai presidenti Berselli e Vizzini siano adeguati rispetto alla propria situazione processuale Lei, oltre ad essere il Presidente del Senato è un autorevole avvocato, come me e come tanti altri presenti in questa sede e sa benissimo, signor Presidente, che un qualsiasi cittadino che sia plurindagato e plurimputato non può scrivere al Senato e veder letta la sua lettera di fronte ai senatori in un'Assemblea che discute di argomenti e di materie che potrebbero riguardare i suoi processi. Lei ci ha letto un testo che alla fine dice: per questo dirò al Consiglio dei ministri - e quindi parla stavolta come Presidente del Consiglio dei ministri - di dare parere favorevole. È lampante il conflitto d'interessi che c'è in questa lettera e siamo fortemente preoccupati, signor Presidente, che lei l'abbia presentata come un atto ufficiale. Un atto di un cittadino che ha problemi con la giustizia, che auguriamo risolva nella sede nella sede competente, ma che non può certo utilizzare la sua funzione istituzionale, mi correggo la sua altissima funzione istituzionale, per cambiare l'ordinamento di questo Paese di fronte a gente che aspetta da anni di vedere giustizia fatta, sia parti lese sia imputati, tutti con uguale diritto, come il nostro ordinamento prevede. Signor Presidente, io sono fra quelli, lo posso dire pubblicamente, che si sono vergognati di aver votato l'indulto. Oggi ci troviamo in una situazione tale che voi potreste porci nella condizione di sospendere i processi: fate un'operazione ancora più pericolosa che è esattamente il contrario del dare giustizia e sicurezza ai cittadini.

atto ad affrontare e a risolvere, sia pure in parte, il grave problema della sicurezza pubblica. Questa opposizione, come è stato riconosciuto dai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, ha contribuito non poco a migliorare il decreto, tanto che i nostri emendamenti sono stati definiti migliorativi. Ora, improvvisamente, ci viene presentata in Aula una richiesta emendativa che con il tema della sicurezza pubblica non credo abbia la benché minima connessione; piuttosto, è connessa fortemente al problema della sicurezza e degli interessi personali del Presidente del Consiglio dei ministri. allora a voi, colleghi della maggioranza, soprattutto a quelli che conosco bene per la loro preparazione, per la loro cultura e sensibilità verso il diritto con la maiuscola, se siete veramente disposti ad appoggiare una riforma di questo genere, che non può che essere definita vergognosa e lesiva dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Signor Presidente, ricordo bene che in apertura di legislatura lei e il presidente Fini avete fatto richiamo alla Costituzione repubblicana ed io fui veramente contento di ascoltare, da parte di uomini che vengono dalla destra, dalla destra, i richiami alla Costituzione. Questo modo di agire lede ed offende i principi della Costituzione, soprattutto quello dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. colleghi della maggioranza: non sottovalutate l'effetto devastante e debilitante per la tenuta morale e politica del Paese. Questo è un messaggio devastante, perché

Presidente, prendo atto che potrò parlare per i due minuti concordati e registro con soddisfazione il fatto che almeno su questo punto lei abbia rivisto quella decisione che consideravo assolutamente non condivisibile, e cioè di comprimere al di là del tollerabile i tempi della discussione. Avuta quindi questa possibilità circoscritta, devo confessare e dichiarare in quest'Aula il mio disagio, il mio imbarazzo e direi anche la mia vergogna in relazione a quello che è accaduto nei giorni scorsi e a come ciò si sta completando qui, adesso. Nelle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali abbiamo discusso con i Presidenti, che vedo in quest'Aula (per la verità vedo il presidente Berselli più interessato al giornale che non a quello che diciamo, ma non importa: evidentemente la questione non ha particolare rilevanza), di una serie di questioni relative ad emendamenti e loro ci hanno dato atto del fatto che alcuni dei nostri emendamenti hanno migliorato il decreto.

e noi abbiamo accettato tutto questo, anche se naturalmente rimanevamo della nostra opinione. Oggi abbiamo questa sorpresa: scopriamo che in Aula si discute di qualcosa che non ha nulla a che fare con il tema del decreto, che non ha nulla a che fare con il tema della sicurezza dei cittadini, ma che ha molto a che fare con la sicurezza di qualche cittadino speciale, che invia lettere al Parlamento e che se le vede leggere; questo è un giorno che sarà ricordato nella storia del Parlamento: è la prima volta che la lettera di un privato cittadino (perché è da privato cittadino che si scrive) viene letta davanti ai parlamentari. È un'offesa al Parlamento e alla Repubblica. Io vi chiedo di ritirare quegli emendamenti, non soltanto che non siano portati al voto; chiedo a voi presentatori di ritirarli perché i nostri lavori in Commissione in seguito possano essere lavori sereni e non ispirati...

Presidente, intendo intervenire ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento e sostenere il non passaggio all'esame degli articoli. Esprimo il mio totale sconcerto e la mia indignazione rispetto alla presentazione da parte dei presidenti, senatore Vizzini e il senatore Berselli, dell'emendamento che sospende i processi. Nella relazione stava scritto che l'obiettivo di questo decreto-legge era quello di accelerare i processi per garantire il diritto di ogni cittadino alla giustizia; questo era l'obiettivo dichiarato e l'esito è un emendamento che sospende i processi. Indignazione e sconcerto che vengono assolutamente aggravati a fronte della lettera del Presidente del Consiglio, un *vulnus* profondissimo al ruolo di questo Senato e al ruolo della Presidenza di questo Senato. Per quello che riguarda la procedura, ritengo assolutamente inammissibile che l'emendamento non sia stato presentato in Commissione e lì discusso, che non sia stato presentato nel testo iniziale, sottoposto alla valutazione della Presidenza della Repubblica, un testo testo assolutamente, peraltro, non pertinente alla materia di cui all'oggetto e pertanto, a mio avviso, da dichiarare assolutamente inammissibile. D'altra parte, proprio ai presidenti Vizzini e Berselli vorrei ricordare quanto hanno argomentato ripetutamente in Commissione, rispetto ad emendamenti che erano stati presentati dal Partito Democratico, in particolare emendamenti che riguardavano la violenza alle donne, lo *stalking*, la violenza ai minori,

Signor Presidente, sinceramente non avrei voluto svolgere questo intervento, perché immaginavo che, viste le reazioni di quest'Aula e letta la lettera del presidente Berlusconi, lei, Presidente, avrebbe ravvisato da sé la necessità di sospendere la seduta e di riunire i Capigruppo.

l'inapplicabilità, se non la contraddittorietà, di queste vostre misure. Sia in Commissione che nelle nostre conversazioni

Paese. Rispetto all'emendamento che il Governo e il presidente Berlusconi ci chiedono adesso di introdurre, quale segnale daremo noi al Paese? Qual è la ragione per cui, per così dire, tutti...

rispetto alla sua sicurezza per introdurre questa norma. È moralmente, prima che costituzionalmente, insopportabile. onorevoli senatori, i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge, ma c'è qualcuno che è più uguale degli altri

secondo gli ordini del Presidente del Consiglio. Noi diciamo che non esiste alcun requisito di necessità e urgenza, come previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Gli emendamenti, signori relatori, configurano una palese violazione dell'articolo 111 della Costituzione, anche in merito ai profili di compatibilità con gli articoli 24 e 25. Badate, sono altre le emergenze del Paese. Qui, all'interno di un decreto, si vanno ad inserire questioni che attengono ad un privato cittadino che vuole risolvere i suoi problemi. Altre sono le emergenze del Paese: il carovita, i mutui che la gente non riesce più a pagare per i cattivi consigli delle banche, la legge sulla *class action* che il Governo si accinge a sospendere, comportandosi da Giano bifronte, perché da una parte il ministro Tremonti, secondo un principio che condividiamo, vuole finalmente far pagare anche coloro che speculano sui *futures*, sui derivati, sul petrolio, dall'altra parte

in virtù di quale alchimia, il vice sindaco di Roma sedeva sui tavoli del Governo? Ma non è questo il tema. L'editto presidenziale che siamo stati costretti ad ascoltare offende la potestà del Senato; contravviene all'articolo 111 della Costituzione, perché inceppa la ragionevole durata dei processi; contravviene all'articolo 25 della Costituzione, perché tende a sottrarre l'imputato al suo giudice naturale; nega il diritto delle parti lese. Tutta la maggioranza si fa sempre bella del fatto che le sue politiche sono a favore delle parti lese: qui c'è una palese e violenta negazione del diritto di tali parti. L'editto presidenziale pretende persino di fissare le udienze e di stabilirne i ruoli e cancella la formazione del libero convincimento del giudice in materia. Assistiamo a qualcosa di inverosimile: il Presidente del Consiglio nella sua lettera afferma che questa è «una situazione che non ha eguali nel mondo occidentale». C'è solo una cosa che non ha eguali nel mondo occidentale: che la televisione sia direttamente al vertice del potere politico e che una persona ineleggibile e incompatibile con l'esercizio del potere politico possa disporre a proprio piacimento delle Assemblee elettive.

per esprimere - e mi piacerebbe che i colleghi ascoltassero - il dramma interiore che sto vivendo oggi: è un atto grave rispetto alla responsabilità della politica. Vengo politica. Vengo dalla lontana Brescia, dalla Val Camonica, e qui, in questa Italia, nata dalla Resistenza e costruita sulle battaglie della verità, si consumano oggi atti che ritengo gravissimi. Voglio vivere ancora in un'Italia libera, forte e democratica. E voglio ascoltare - lo dico fin da ora agli amici della Lega Nord - con grande con grande attenzione e grande responsabilità la loro riflessione su questo tema, perché non credo che quella parte politica così importante oggi nel tessuto sociale del Paese la pensi in questo modo. Mi richiamo, dunque, all'articolo 96 del Regolamento del Senato

modifica proposta nella giornata di ieri dai relatori non risponde in alcun modo ai requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. L'Aula non ha titolo, ad avviso dell'Italia dei Valori, per pronunciarsi sulla sussistenza di tali requisiti e quindi per procedere all'esame del disegno di legge di conversione, inserendo nel decreto-legge le norme in questione, senza valutarne la rispondenza con il citato articolo 77 e determinando così un vizio *in procedendo,* come ribadito da ultimo nella sentenza n. 128 del 2008 della Corte costituzionale.

ascoltate le parole che Silvio Berlusconi - non è chiaro se come Presidente del Consiglio o come cittadino imputato - ha rivolto a lei e per suo tramite a quest'Aula, è difficile sfuggire al dubbio che tutto il gran parlare che il Governo ha fatto e sta facendo sulla necessità e l'urgenza di occuparsi di sicurezza, di lotta all'immigrazione clandestina, di difesa della *privacy* dei cittadini sia il pretesto per altre necessità e urgenze: quelle personali del Presidente del Consiglio.

La motivazione principale che viene addotta è la mancanza di ogni certezza del diritto e di affidabilità da parte di un Paese che non solo non rispetta le regole, ma ha dieci milioni di processi pendenti, quattro milioni dei quali di natura amministrativa, che riguardano l'economia. Come possiamo pensare di dare sicurezza ai nostri cittadini impedendo l'esecuzione dei processi? Come possiamo pensare che la sicurezza sia un tema

Presidente, anch'io nutro sgomento, come tanti altri colleghi. La lettera è stata letta a mezzogiorno. Un famoso romanzo di tanti anni fa "Buio a mezzogiorno". di una gravità inaudita. Faccio un'ulteriore considerazione: talvolta un episodio si incarica di dare l'idea più di tanti discorsi dello stato dell'arte. Questo episodio ci ha dato esattamente l'idea di quella cosa che non volevamo chiamare «rischio di regime» e che da oggi siamo costretti a definire tale. Mi auguro che le colleghe e i colleghi

valga la pena di rompere una prospettiva di dialogo nel rispetto dei ruoli tra maggioranza ed opposizione ponendosi insieme davanti ai problemi dell'Italia e riportare nel Paese il clima di scontro frontale dal quale stavamo uscendo. Ne vale la pena, onorevoli colleghi? L'Italia non avrebbe diritto ad avere una classe dirigente e di governo capace di volare alto? Vi chiedo, colleghi presentatori, ne vale la pena? E per che cosa?

Lo sa il Presidente del Consiglio che noi non siamo il suo collegio di difesa, che quest'Aula non è un'aula di giustizia, ma è un'Aula del Parlamento? Noi non siamo qui - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del centrodestra - per sostenere un provvedimento *ad personam*, non siamo qui per studiare una strategia processuale a favore del Presidente del Consiglio: siamo qui perché siamo stati eletti dai cittadini ed è ai cittadini - a tutti i cittadini e non al Presidente del Consiglio - che dobbiamo rispondere. L'Italia dei Valori ha capito sin da subito che l'apertura al dialogo avviata dal Presidente del Consiglio all'inizio della legislatura era semplicemente una rappresentazione teatrale. Come ha detto il direttore Scalfari, che mi permetto di citare in quest'Aula, «il Presidente del Consiglio sta recitando il ruolo di uno statista». Per tale motivo noi dell'Italia dei Valori siamo stati fin dall'inizio vigili sui provvedimenti del Governo, e bene abbiamo fatto. Onorevoli colleghi del centrodestra, vi sollecito ad avere un moto di orgoglio e a riconoscere che l'emendamento che sospende i processi è inaccettabile

Signor Presidente, facendo riferimento anche al suo discorso di insediamento, voglio credere ed auspicare che saprà mantenere, nel corso della direzione dei lavori di questa Assemblea,

pubblica lei saprà accogliere la richiesta avanzata più volte di una convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo. D'altra parte, la lettura della lettera del Presidente del Consiglio dimostra con chiarezza che

i processi per decreto, e - guarda caso - questa sospensione riguarda anche il Presidente del Consiglio. È gravissima e scandalosa anche per le modalità una lettera che tutti abbiamo potuto ascoltare, con la quale il Presidente del Consiglio intima al Senato di procedere speditamente sulla base delle indicazioni dei suoi legali. Ripeto, questo è un atto assolutamente vergognoso! Ed è del tutto evidente, signor Presidente...

e soprattutto con la lettera del Presidente del Consiglio, stiamo stravolgendo il nostro sistema di garanzie e il nostro sistema democratico e stiamo mettendo a repentaglio l'immagine del nostro Paese nel mondo e in Europa,

la Santa Sede e il Papa, ho avuto un sussulto e da repubblicana e democratica mi sono chiesta se la forma di questo Stato sia ancora repubblicana o se nella sostanza non si stia trasformando decisamente in una struttura monarchica. Oggi il delirio di onnipotenza, forse benedetto anche dalle gerarchie ecclesiastiche interessate, è andato oltre, con un'incursione selvaggia in questo decreto, in cui si confonde l'interesse del popolo italiano con l'interesse personale. personale. Questo mette in seria difficoltà noi e anche lei, Presidente, perché - vogliamo ricordarlo al Presidente del Consiglio - ancora rappresentiamo il popolo italiano, la sua sicurezza, i suoi interessi e non quelli della Sua persona, ancorché lui si creda l'onnipotente.

che prefigura un diritto in testa a ciascun senatore, non sia interpretabile con l'applicazione del comma 5 dell'articolo 55, che determina i tempi da assegnare ai singoli Il comma 1 dell'articolo 96 stabilisce che ciascun senatore - quindi 315 senatori - può esercitare il medesimo diritto. Lei non può precludere

Noi dobbiamo affrontare temi nuovi, che sono stati introdotti anche dalla lettera del Presidente del Consiglio. Ringraziamo lei, presidente Schifani, per avercela letta, ma vogliamo che il Presidente del Consiglio comunichi al Senato, con la sua presenza, le sue osservazioni e le sue pretese in ordine ai disegni di legge. Lei

Signor Presidente*,* lo slogan del Popolo della Libertà durante la campagna elettorale recitava: «Rialzati, Italia! Il Governo Prodi ti ha messo in ginocchio». Le emergenze che si elencavano erano soprattutto la sicurezza, i rifiuti in Campania, le condizioni precarie delle famiglie italiane. Invece, tra i primi provvedimenti il Governo ha pensato subito a salvaguardare Retequattro e, anziché affrontare con attenzione i rischi, le insicurezze, le preoccupazioni che i cittadini vivono davvero quotidianamente e porvi rimedio, oggi, con il pacchetto sicurezza, si passa a cancellare con un colpo di spugna i processi per chi attende giustizia - mi ripeto, perché è stato già detto dai miei colleghi per agevolare soltanto il Presidente del Consiglio. Siamo davvero sconcertati. Torniamo alle leggi *ad personam*. Questo è inaccettabile. È un oltraggio alla nostra Costituzione, a quanti hanno sacrificato la loro vita per un Paese democratico. A tutti gli onorevoli colleghi del centrodestra dico oggi: svegliatevi! Aprite voi gli occhi! Salvaguardiamo la nostra Repubblica da una strisciante dittatura che ci renderà alla pari, purtroppo, dei Paesi del Terzo mondo.

della discussione, della nuova impalcatura del decreto-legge è l'emendamento di cui stiamo discutendo, credo che sarebbe sufficiente modificare il titolo del decreto-legge n.

dall'automatismo dell'espulsione all'aggravante comune, al nuovo reato di cessione a titolo oneroso di un immobile a cittadini non in posizione regolare. Adesso aggiungiamo

Credo che su questo affossamento dello Stato di diritto e dei principi della Corte costituzionale aveva visto giusto

saggio e di dare retta al Presidente del Consiglio che vuole risolvere i problemi e non complicarli. È vero, Sottosegretario, vuole risolvere i problemi suoi. Noi dell'Italia dei Valori lo aiuteremo a complicarli.

Signor Presidente, oggi lei ha chiesto un minuto di raccoglimento per le morti degli immigrati nel canale di Sicilia. Quando una donna incinta con due bambini affronta il mare forza 5 o 6 non lo fa per venire a delinquere, ma perché ha fame. Nella maggioranza, nonostante il minuto di silenzio, qualche forza politica la pensa diversamente e vorrebbe la Marina attivarsi per applicare regole di ingaggio violente contro i barconi. Ma come mai, invece, sulla vicenda in questione in nessuno di voi emerge un sentimento di indignazione per la lettera inviata dal Presidente del Consiglio che parla delle indicazioni dei suoi avvocati? I relatori che presentano questo emendamento non provano nulla? Siamo di fronte ad un golpe bianco da parte di colui che ha vinto le elezioni, che ha nominato gli eletti che difendono lo scranno, ma non la propria coscienza. In Parlamento qualcuno si assunse la responsabilità politica dell'omicidio dell'onorevole Matteotti. Altri tempi. Questo è uno Stato che nasce dalla Resistenza. Avete vinto, ma non macchiatevi di questo torto allo Stato e all'Aula. Non parlate alle carceri, parlate agli italiani. E tu, Renato Schifani, non sei qui l'amico di Silvio Berlusconi. Ma lei...

siano incostituzionali anche per violazione dell'articolo 111 della Costituzione sulla durata ragionevole del processo. Vi invito dunque a ritirarli, perché parti offese e imputati hanno il diritto di veder conclusi i loro processi indipendentemente da quello che riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri.

una cosa che nessuno ha ascoltato. Vorrei che rileggesse di nuovo il suo intervento per iniziare poi il dibattito, magari nel pomeriggio. È nostro diritto capire che cosa egli ha detto. Presidente, le chiedo di riconsiderare la decisione che ci ha comunicato poco fa, in base alla quale, benché ci siano diversi colleghi che hanno chiesto

Questi due principi non possono che essere contemperati e applicati entrambi e quindi è evidente che il diritto di ciascun senatore di proporre tale questione nei termini in cui ciò è riconosciuto dal Regolamento deve prevalere su una decisione della Conferenza dei Capigruppo. Pertanto, le chiedo di consentire lo svolgimento di tutti gli interventi a partire dalla seduta pomeridiana e poi di passare al voto.

parlare prima del voto, così come questa Presidenza non impedirà mai a ciascun Capogruppo di maggioranza o di opposizione di poter intervenire quando lo riterrà opportuno.

«che dovrebbe far riflettere i colleghi del centrosinistra, che si sia introdotto di soppiatto, di nascosto in un decreto-legge un nuovo reato che nulla ha a che vedere con questa tematica». Poi proseguiva dicendo: «Ci riserviamo di assumere iniziative serie, perché non si può continuare ad accettare questo andamento dei lavori, che non può essere tollerato nemmeno da parte della Presidenza» - allora presiedeva il senatore Marini - «senza un sussulto di dignità e ci appelliamo anche con rispetto al Capo dello Stato che vigila sull'andamento delle nostre istituzioni. Non si può continuare ad accettare che si metta in votazione un emendamento che introduce un nuovo reato su temi che toccano la sensibilità e la coscienza dei cattolici» - allora erano i cattolici, mentre oggi la platea è molto vasta e riguarda tutti i cittadini italiani - «proprio in un decreto che nulla ha a che spartire con questa tematica. Tra l'altro, l'argomento non era mai stato portato all'attenzione della Commissione competente e dell'Aula perché non esisteva alcun emendamento posto all'esame della Commissione e dell'Aula». Potrei continuare, ma non voglio abusare della sua pazienza. Signor Presidente, credo che se volessimo dare continuità ai nostri lavori e fossimo tutti coerenti